Signora Presidente, signori del Governo, colleghi del Senato, come ho già detto ieri, quando ho commentato la richiesta del Governo di porre la questione di fiducia su questo testo legislativo, che la storia di questo provvedimento è cominciata male ed è finita peggio. Infatti, il vizio originario di quest'atto, al di là del suo contenuto, è il modo opaco, quasi fraudolento, per quanto formalmente corretto, con cui è stato posto all'ordine del giorno del Senato. Si tratta del classico caso in cui il formalismo giuridico fa torto alla sostanza, con un'interpretazione regolamentare ineccepibile, che viene però percepita come ingiusta. Il Presidente del Senato, con qualche imbarazzo, ben consapevole di questo tarlo originario, che corrodeva la vita stessa del provvedimento, ha provato a ricondurlo ai canoni di una corretta dialettica parlamentare, ma l'ultimo atto del Governo - quello di porre in modo ingiustificato la questione di fiducia - ha reso inutile anche questo tentativo. E proprio il *modus agendi* non ha fatto che inasprire gli animi e le posizioni delle parti politiche, già improntate a dura contrapposizione. Peraltro, non ci ha stupito la natura di questo disegno di legge, perché, in fin dei conti, quest'iniziativa legislativa ben si inserisce nel solco - anzi, nella prassi ormai consolidata - di quei numerosi interventi in materia di giustizia che si usa definire leggi *ad personam*, dispositivi che si caratterizzano per l'assenza di un interesse generale e che forse faremmo bene a non chiamare più leggi, dal momento che la norma è tale quando sussistono i requisiti di generalità e astrattezza. Invece, questi provvedimenti nascono al fine esclusivo di intervenire - o peggio, di interferire - nei procedimenti che vedono interessato il *Premier* e i suoi più cari amici. Si è resa infatti sempre più evidente un'anomalia, tanto eccezionale quanto pericolosa, che contraddistingue questo Governo e la sua maggioranza, tale per cui la salvaguardia dell'incolumità processuale del *Premier* ha assunto ormai rango di funzione costitutiva, da cui dipende la stabilità dell'Esecutivo e la tenuta politica dell'accordo di maggioranza. In questi giorni, nell'Aula del Senato, molti interventi - alcuni dei quali pregevolissimi, anche dal punto di vista tecnico - ci hanno illustrato tutti i limiti, le debolezze e le contraddizioni di questo provvedimento, nonché i più gravi effetti distorsivi determinati da questa sequenza di provvedimenti che, con foga quasi compulsiva, sono stati predisposti per tentare di risolvere - in modo quasi sempre inefficace - i troppi problemi giudiziari del Presidente del Consiglio. Ed è anche il precipitato di queste iniziative infelici in materia di giustizia - ormai del tutto estraneo al sentimento profondo del Paese, come dimostrato dall'esito del *referendum* sul legittimo impedimento a restituirci il dato più autentico di questa stagione politica, che è il completo fallimento di questo Governo. È un fallimento eclatante, che prende sostanza proprio a partire dalla mancata riforma della giustizia, tanto annunciata quanto mai davvero affrontata. Si sono preferiti infatti interventi parcellizzati, spesso dannosi, i cui effetti concreti non hanno prodotto altro che l'indebolimento di un pilastro fondamentale delle funzioni essenziali dello Stato. Infatti, anche in questo caso il combinato disposto tra questo provvedimento e i termini di prescrizione ridotti che derivano dal processo breve determina la sostanziale impossibilità di celebrare molti processi e quindi di emettere sentenze e di comminare pene, producendo di fatto l'esito di una denegata giustizia. A conferma ulteriore della non credibilità di questo Governo in materia di politiche sulla giustizia, basta ricordare l'enfasi con la quale nel marzo scorso fu annunciata l'ennesima epocale riforma di sistema, accompagnata dalla rassicurazione che mai più vi sarebbero stati interventi legislativi per provvedimenti *ad personam*. Quando il presidente del Consiglio Berlusconi dava questo annuncio solenne, sedeva accanto a lui il ministro guardasigilli Alfano: speriamo che l'impegno del nuovo segretario del Popolo della Libertà di dare vita ad un partito di onesti non abbia la stessa coerenza logica che ebbe quell'impegno sulle leggi *ad personam.* Voglio dire che questa linea ha sprecato tante possibilità di dialogo e di apertura di confronti politici, perché quando quella posizione fu annunciata dal Presidente del Consiglio l'area politica che si definisce Terzo Polo dichiarò la propria disponibilità al confronto parlamentare sul tema della riforma della giustizia, che è un'esigenza dell'intero Paese. Ma la linea di comportamento che anche oggi confermate ha reso impraticabile quello spazio di dialogo che era stato annunciato. Quello che spiace constatare anche oggi è che il recentissimo insediamento del nuovo Ministro della giustizia - al quale rivolgiamo comunque un augurio di buon lavoro, e ne ha davvero bisogno, vista la delicatezza del suo incarico - malgrado le sue prime positive dichiarazioni è stato accompagnato dall'improvvida iniziativa del Governo di porre la questione di fiducia su questo provvedimento. Solo che, mentre il Governo chiede la fiducia al Parlamento su questo atto, è il Paese che revoca la fiducia a questo Esecutivo, incapace ormai di affrontare le vere questioni su cui si decide il destino della Nazione in un momento tanto delicato. Questo atto viene compiuto oggi nel momento storico in cui la nostra economia è sotto attacco ed è un altro passo verso la inevitabile fine di quest'esperienza politica. Speriamo non sia un passo verso il baratro per il Paese. Tra l'altro, questo passaggio politico si pone in aperta contraddizione, compromettendone forse in modo irrimediabile le prospettive virtuose, con l'azione saggia del Capo dello Stato, il quale solo poche ore fa ha rivolto alle forze politiche il rinnovato invito di procedere su un percorso di riforme condiviso anche in materia di giustizia. La costruttiva opera del Presidente della Repubblica ha determinato per un momento le condizioni per un clima di collaborazione istituzionale che, pur nella doverosa distinzione delle responsabilità dei ruoli tra maggioranza e opposizione, ha ha permesso di garantire credibilità alle istituzioni del nostro Paese in un momento difficile e, di fatto, ha favorito maggiore efficacia alla stessa azione di governo, come è avvenuto con la eccezionale velocità di approvazione della manovra di stabilità finanziaria di poche settimane fa. A fronte di questa azione così autorevole, c'è un Governo che passa da iniziative estemporanee e propagandistiche, se non vogliamo considerarle destabilizzanti, come quella di aprire sedi ministeriali nella Villa Reale di Monza, che costringono il supremo garante dell'unità nazionale a censurare formalmente questi atti, alla prepotenza di imporre al Parlamento l'approvazione a tappe forzate di una legge *ad personam* tra le più dannose per la funzionalità del nostro sistema giurisdizionale. Senza voler evocare altre ulteriori gravissime questioni, è evidente a tutti come questa maggioranza non sia più in sintonia con il Paese e quindi in grado di garantirne gli interessi fondamentali in questa fase così drammatica. Anzi, con la sua azione accentua ogni giorno di più il distacco tra i cittadini e le istituzioni repubblicane, alimentando maggiormente quel sentimento di livore e di avversione per gli istituti della democrazia rappresentativa che, con linguaggio gergale, definiamo antipolitica. Se i rappresentanti di questo Governo avessero piena consapevolezza delle loro responsabilità istituzionali, non potrebbero più sottrarsi al dovere inderogabile di lasciare ad altri la guida del Paese; ma, chiusi come sono nel circuito perverso del loro personale destino, non sono in grado di comprendere ciò che è giusto e doveroso nell'interesse della Repubblica. Per queste ragioni, con piena convinzione, votiamo no al provvedimento e neghiamo la fiducia al Governo.

Mentre l'Italia è alle prese con enormi difficoltà nel collocamento del proprio debito, mentre la Germania disinveste dal nostro Paese, mentre indagini e inchieste della magistratura aprono squarci inquietanti su importanti settori industriali ed economici delle maggiori imprese pubbliche, al punto da legittimare voci sempre più insistenti di prossime dimissioni - non solo da inquilino - del potente Ministro dell'economia, mentre non si riesce ad agganciare un qualsiasi *trend* di crescita decente, in particolare a causa dell'ormai inesistente livello di credibilità raggiunto dal Governo attuale, mentre le parti sociali ci chiedono discontinuità e l'opinione pubblica mostra tutto il suo distacco nei confronti delle istituzioni, mentre accade tutto ciò, l'agenda politica imposta dalla maggioranza e dal Governo, invece di concentrarsi sulle emergenze del Paese, costringe tutti ad inseguire bizzarre dislocazioni di sedi ministeriali, oppure non trova altro di meglio da fare che tenere inchiodato il Senato della Repubblica a discutere e a votare una fiducia su di un provvedimento di cui, sinceramente, per come è venuto configurandosi, nessuno sentiva la mancanza. Eppure, come ha già giustamente sottolineato il presidente Rutelli qualche seduta fa, le opposizioni, sostanzialmente, nel loro complesso, hanno già avuto modo di dimostrare una disponibilità a farsi carico della delicata situazione del Paese, sia nella fase di approvazione della manovra economica che nel passaggio in Aula del rifinanziamento delle missioni militari. Noialtri abbiamo scelto la strada della responsabilità verso il Paese, e pensavamo che sareste stati in grado di cogliere questa nostra disponibilità. Invece, dobbiamo registrare che proprio non vi rendete conto dei rischi che stiamo correndo, e anzi vi ostinate a percorrere, ancora una volta, i soliti sentieri dello scontro frontale, consapevoli che a nulla porteranno. E ci dispiace veder sciupare in questo modo occasioni importanti: infatti, non possiamo non sottolineare anche noi il rammarico che abbiamo provato nel verificare la distanza siderale tra le dichiarazioni che hanno accompagnato la nomina del neo Guardasigilli e la procedura di richiesta della fiducia messa sul provvedimento che stiamo esaminando Ma, signor Ministro, è in questo modo che pensa di stimolare un confronto maggiormente sereno sulla giustizia? Dica una parola su questo provvedimento! Eppure noi, formalmente, stiamo discutendo di un provvedimento nato su iniziativa parlamentare, e non governativo; un disegno di legge che avrebbe dovuto riguardare l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Peccato che nel frattempo ci troviamo di fronte a tutt'altro! Una sorta di "fine dibattimento mai". Un atto ampiamente rimaneggiato in Commissione, che va oltre ogni intenzione dei proponenti. Questo provvedimento doveva essere in verità una bandiera, più simbolica che sostanziale, della Lega e di quelli a cui piace mostrare la "faccia feroce" all'opinione pubblica. Ma, per come era congegnato, sinceramente avrebbe potuto stimolare una reale discussione politica e parlamentare su almeno due questioni importanti. La prima verte sull'utilizzo del giudizio abbreviato e alla sua utilità. Infatti è ormai abbastanza evidente come sia venuto meno l'obiettivo deflattivo insito nell'introduzione del rito abbreviato e, soprattutto, come i benefìci ad esso connessi siano utilizzati solo allorquando si restringono in maniera significativa tutti gli altri spazi difensivi. Si poteva discutere di questo oppure ci si poteva confrontare su un altro tema che - a mio avviso - pone questioni di legittimità costituzionale, investendo gli articoli 3, 27 e 111 della Costituzione. lo sono tra quelli che non sono affatto convinti che affidare alla pena, quantunque legata a reati ignobili, solo caratteri afflittivi e non anche di rieducazione della persona sia un reale avanzamento sul piano della civiltà giuridica. Capisco che si tratta di un confronto delicato tra diverse sensibilità culturali e politiche sul tema del "fine pena mai". Nel dibattito di ieri in Aula ho avuto modo di richiamare il pensiero di Aldo Moro quando diceva che «per quanto riguarda il come debba essere una pena, debba essere dato in linea di principio un giudizio negativo non soltanto per la pena capitale (...) ma anche nei confronti dell'ergastolo». Ma capisco che si trattava di altri tempi. Magari c'era pure il proporzionale, non c'era il sistema bipolare: tuttavia, allora la discussione sulla giustizia aveva altro spessore, e il rispetto delle istituzioni impediva che si potessero piegare con tanta supponenza delicati equilibri costituzionali agli interessi di singoli individui. Purtroppo, però, non si è potuto né si è voluto discutere di tutto questo. Questo provvedimento (stravolto da un emendamento che nessuno riesce a spiegare perché non sia stato dichiarato inammissibile) ha costretto quelli della "faccia feroce" a diventare distratti, a piegarsi e a girarsi dall'altra parte appena sono tornati preminenti gli interessi giudiziari La verità è che sul testo licenziato dalla Camera dei deputati, o sullo stesso testo originario, non si sarebbe mai posta la questione di fiducia. L'emendamento si è mangiato il testo originario e l'ha digerito. E noi votiamo la fiducia non più sull'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo ma sul "processo lungo". E pensare che vi erano anche questioni sull'emendamento che si potevano discutere con serenità! Niente da fare. Avete un solo obiettivo: tutelare sempre e solo l'interesse processuale del Presidente del Consiglio. Per questo avete introdotto la procedura del "fine dibattimento mai", attraverso la puntualizzazione della facoltà di far interrogare testimoni chiamati dalla difesa senza alcun limite. Ma avete riflettuto veramente che, oltre ai processi in cui è coinvolto il *Premier*, ve ne sono altri? Provate ad immaginare cosa può accadere quando lo stupratore, il capo della cosca, lo 'ndranghetista, il mafioso potrà guardare negli occhi il testimone che sta interrogando durante il processo. È proprio per tale questione che pensiamo che abbia ragione da vendere il CSM, quando segnala che si rischia concretamente di rallentare tutti i processi penali in corso, a parte quelli per i quali si è chiuso il primo grado. E ha ragione da vendere l'ANM, quando denuncia la devastazione del processo penale. La verità è che ci avete raccontato che il processo breve era la più importante riforma di tutte le riforme della giustizia italiana, un fatto indispensabile per riportare i tempi del processo italiano nella media europea. Adesso volete propinare agli italiani che il processo lungo, e quindi la possibilità per l'imputato di chiamare a testimoniare quante persone vuole senza che il giudice possa realmente opporsi, è un fatto di civiltà giuridica. Di sicuro non potete non comprendere come l'effetto combinato dei due dispositivi confermi tutte le preoccupazioni segnalate. io credo che questa fiducia sia un evidente ed ulteriore segno di debolezza del Governo. Questo è un Governo ormai logorato, che è minoranza nel Paese e nell'opinione pubblica e che, non avendo più il consenso reale, si trova tristemente condannato a tenersi in vita appoggiandosi a sistemi di quel teatrino della politica tanto criticato proprio da Berlusconi. Siete costretti a fare un Ministro ogni mese e un Sottosegretario ogni settimana. Siete sotto ricatto politico interno e commissariati in Europa, siete senza una comune politica estera, dovete marcarvi a vista anche nel modo come portate i provvedimenti nel Parlamento o nel Consiglio dei ministri: un Ministero a Monza a te, una norma sull'immigrazione a te, una leggina aggiusta-processi a me. Non può più continuare in questo modo. Il Paese ha bisogno di un Governo che abbia un sostegno ampio, amplissimo. Ha bisogno di una fase in cui si affrontino unitariamente le riforme indispensabili, comprese quelle della giustizia, sulle quali è naufragato il bipolarismo italiano. Il Paese ha necessità di ritrovare fiducia in se stesso e in una rappresentanza istituzionale e politica che sappia raccogliere l'invito che ci giunge dal Capo dello Stato, e che possa superare questo ventennio di promesse mancate e di obiettivi falliti. Anche per questo, noi del Terzo Polo voteremo contro la fiducia, nella consapevolezza che non avete più la maggioranza nel Paese e che prima trovate in voi stessi la forza di licenziare questo Governo, prima si potrà aprire una nuova stagione di responsabilità, che sappia unire tutti gli italiani,

l'articolo 161 del Regolamento, che introduce l'istituto della fiducia, è corredato dai pareri della Giunta Il più importante parere della Giunta, che ha interpretato l'articolo 161, ha fissato questo principio: la rilevanza costituzionale della discussione sulla fiducia assume carattere preminente, avendo il Governo condizionato in modo espresso all'approvazione di un testo la propria sopravvivenza. In questa formula della vostra parabola, avete cominciato negli otto dei nove anni degli ultimi undici di vostro governo, con le rogatorie, il falso in bilancio, il legittimo sospetto,

"processo breve" per determinare la morte dei processi per prescrizione e ora il "processo lungo". Voi avete sbagliato sempre, senza commettere errori: ed è veramente una condizione unica, quando si riesce a sbagliare sempre senza neanche incorrere nell'errore di fare qualcosa di giusto. Si sbaglia sempre. Ed è una falsificazione quella di dire che siete stati costretti a porre il voto di fiducia per contrastare l'ostruzionismo dell'opposizione. Avete posto il voto di fiducia dopo circa tre‑quattro ore di discussione, ed era talmente ostruzionistica la nostra opposizione che, grazie alle nostre ripetute, alcune volte urlate, sollecitazioni avete parzialmente modificato il testo, recependo alcune delle nostre critiche: altro che ostruzione! Se fosse proseguita la discussione, probabilmente altre altre nostre sollecitazioni sarebbero state recepite. Così come dovete finirla con i falsi comiziali: andate nelle borgate a fare i comizi! *(Applausi dal Gruppo voi dovete rispettare, rispettare, rispettare! Voi dovete rispetto!

perché il testo che voi avevate proposto era una cambiale da onorare da parte di qualcuno alla mafia. Voi siete espressione della decadenza di un potere arrogante, concentrato sulla protezione del capo assoluto; non vi interessano i cittadini. Per anni avete rinunziato al richiamo della coscienza. Voi siete ormai i berlusconiani, ossia l'espressione del berlusconismo, che è la malattia del Paese. Molti di voi, dobbiamo riconoscerlo, provano vergogna. Molti di voi hanno da tempo perso anche la capacità di vergognarsi. Il servilismo, antico male italiano, ha intaccato la mente. Il corpo della politica è invaso dalle metastasi. Voi siete la causa della montante antipolitica, avvilendo il Parlamento, che è visto come il male assoluto. Voi non avete giustificazioni, non potete inventarvene. Voi avete fatto un capolavoro di strafalcioni giuridici,

sappia l'Aula, la nostra disponibilità a consentirvi di cambiare il testo su cui avete posto la fiducia, con disprezzo assoluto del Regolamento. Si voleva cioè porre la fiducia su un altro testo e si chiedeva la nostra complicità, perché sapevate che questo testo sarà inesorabilmente bocciato anche dagli studenti dai Gruppi IdV e PD)*. La vostra concezione della democrazia parlamentare è marcia e vergognosa; la vergogna però è tutta vostra, perché voi ne siete la causa. Ed onde evitare disinformazione, avendone alcuni giornali parlato, è bene fare chiarezza: quando ieri, quando ieri, per un gesto di stima che confermo, ho fatto presente al sottosegretario Caliendo che nel corso del mio intervento avrei sottolineato gli strafalcioni giuridici, è altrettanto vero che, con la sua onestà, il sottosegretario Caliendo mi ha chiesto la disponibilità a cambiare il testo. Io risposi ieri che non potevo rinunciare al mio intervento in Aula, e che un'eventuale sua richiesta non poteva essere fatta in un'Aula semideserta, ma doveva essere fatta in un'Aula come quella questa mattina, ad esempio. È altresì vero che i funzionari del Senato hanno avvertito che una cosa del genere non poteva farsi e che mai si era fatta. Ma voi volevate farla. I cittadini ci guardano e giudicano. Voi non siete capaci di governare neanche a colpi di fiducia: sbagliate pure quando ponete la fiducia! Noi dobbiamo salvare le istituzioni dal discredito e dalla rabbia montante del popolo italiano. Avete troppo presto dimenticato i *referendum*; avete dimenticato quel maldestro tentativo di cambiare la legge sul nucleare sei giorni prima del voto. Ci avete provato sempre, vi hanno detto di no e siete stati sommersi dal voto degli italiani. Quanto ancora volete resistere? Quanto ancora resisterete al fango ed alla cattiva coscienza che vi soffoca? Ora darete la fiducia, ma ne sarete travolti, paradossalmente: più cercate la fiducia per scappare dal Parlamento, più affondate nella sfiducia del popolo italiano. Arroccati in un potere che si sgretola, voi sarete ricordati come la pagina buia della democrazia. Siete assediati dall'esterno e vi assediate vicendevolmente. Ora fiduciatevi, e annunciate al popolo la buona novella. Quando finirete non avrete perso solo la rappresentanza politica, ma sarete costretti a provare a recuperare la vostra dignità. Voi non cadrete in piedi, ma con le spalle al popolo, inciampando nel tentativo di scappare e cercando di evitare i meritati e sacrosanti calci nel sedere.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, è vero quanto hanno affermato molti colleghi dell'opposizione: questo disegno di legge ha rappresentato l'occasione per modificare previsioni, processuali e non, diverse rispetto all'impianto originario. Tuttavia, è noto a chi frequenta le Aule parlamentari e non si nasconde dietro il velo dell'ipocrisia come sia più facile effettuare tanti piccoli aggiustamenti rispetto a riforme monumentali. L'occasione è stata utilizzata per correggere storture del sistema non più tollerabili, mantenendo, seppure sotto altra forma, il principio originario della legge. Non è possibile concedere uno sconto automatico di pena a chi va condannato alla pena massima del nostro ordinamento, l'ergastolo, essendosi macchiato dei peggiori delitti solo perché ricorre al giudizio immediato. L'occasione è stata utilizzata per ottenere un processo più garantista, attuando una sostanziale *par condicio* probatoria tra accusa e difesa, ma anche per rendere più certa l'espiazione in carcere della pena ed evitare che pericolosi criminali godano di benefici troppo presto, con il rischio di un ritorno troppo anticipato al crimine. Un processo più garantito nella prova, perché basata su un presupposto oggettivo, la pertinenza, facilmente riscontrabile mediante un giudizio *ex ante* da parte del giudice, in virtù del legame tra il teste e l'evento o il comportamento da provare. Non la rilevanza o la non superfluità, dunque, tipici di una valutazione possibile solo *ex post*, dopo l'assunzione della prova, e non *ex ante*, come richiesto oggi al giudice. Come può fare un giudice a ritenere rilevanti o non superflue delle dichiarazioni, se prima non le ha sentite? ha sentite? In tutto ciò c'è il rischio di un giudizio presuntivo o superficiale, spesso largamente discrezionale e, in molti casi - eccellenti e non - puramente arbitrario. Alcuni colleghi si sono affidati all'iperbole per criticare la riforma, dimenticando la possibilità per il giudice di escludere le testimonianze manifestamente sovrabbondanti, ancorché pertinenti in astratto (articolo 468 del codice di procedura penale), di revocare i testi ammessi in corso istruzione dibattimentale, risultando superflui e manifestamente non pertinenti. C'è poi chi ha spolverato rischi per l'antimafia, rievocando eventi tragici. Questa maggioranza e questo Governo non temono critiche al riguardo, avendo segnato veri e propri *record* nella lotta alla mafia e al terrorismo, sul campo e nelle Aule parlamentari.

per significare a chiare lettere l'impossibilità di riascoltare dichiarazioni alla base di motivazioni di sentenze per tali reati acquisite agli atti di altro processo, per rimettere cioè in discussione sentenze sull'associazione mafiosa. Dispiace che molti colleghi autorevoli del centrosinistra abbiano sacrificato la loro credibilità sull'altare della demagogia, ritenendo possibile che l'imputato possa interrogare direttamente:

rappresentando comunque un campione pericolosamente incline ad esegesi abnormi, riscontrabile, per fortuna in modo isolato, anche in magistratura. Dispiace, infine, l'ostruzionismo nei confronti dei limiti formulati ad una legge Gozzini, interpretata troppo di frequente con superficiale disinvoltura e buonismo da alcuni magistrati, all'origine di gravi delitti perpetrati proprio da pericolosi criminali, che avrebbero dovuto rimanere più tempo nelle nelle patrie galere. Ma da che parte state? Siete con i cittadini, che tremano e si indignano, rivedendo dopo pochi anni sotto casa omicidi e sequestratori, o siete con i magistrati che vogliono ancora mantenere il privilegio della discrezionalità incolpevole? Voi del centrosinistra invocate le grandi riforme, dichiarandovi pronti a collaborare con la maggioranza per migliorare il «pianeta giustizia», ma non vi scandalizzate se il pubblico ministero richiede il giudizio immediato e poi presenta una lista di 130 testimoni: in questo caso niente processo lungo? Immaginate se lo avesse fatto la difesa! È stato poi fatto il solito elenco di leggi *ad personam*: ma perché non le avete abrogate nella scorsa legislatura? Bastava un tratto di penna, un decreto-legge. La verità è che continuate a voler perseguire la via giudiziaria per abbattere l'avversario politico. La verità è che l'antiberlusconismo per voi è ragione di vita politica: in assenza di capacità di suscitare consensi con ricette politiche, continuate a suonare sempre la stessa musica.

perché eravate sotto attacco da parte di quei magistrati chiamati oggi alla guerra santa contro Berlusconi; i soliti crociati,

in quanto sono gli unici portatori della verità. In quella legislatura, fu modificato il reato di abuso d'ufficio, con una legge *ad personas*, in quanto troppi vostri personaggi eccellenti rischiavano grosso. Se volete realizzare il dialogo e la condivisione più volte invocati dal Presidente della Repubblica, abbiate il coraggio di abbandonare i legami che vi hanno impedito finora anche solo di sedervi a discutere. Noi le riforme le abbiamo messe in cantiere e in parte realizzate. Perderemo eventualmente le elezioni, ma non sarete certamente voi a vincerle, perché non avete programmi: c'è il vuoto pneumatico nel vostro schieramento, sapete solo colpire, insultare, offendere, senza proporre qualcosa di alternativo. Perderemo quella voglia di rinnovamento alla base del consenso espresso al centrodestra dagli italiani, quella voglia di perequazione tra Nord e Sud, di sburocratizzazione, quella voglia di un sistema pubblico snello, rapido ed efficiente, quella voglia di maggiore tutela dei più deboli e dei meno abbienti. Noi proseguiremo in questo cammino, meglio se con voi, ma anche senza. Per queste ragioni, il Gruppo Coesione Nazionale-Io Sud‑Forza del Sud voterà la fiducia a questo Governo.

votiamo no alla fiducia, e votiamo contro questo provvedimento, perché - come sempre accade quando vi occupate di giustizia - trasformate provvedimenti giusti in provvedimenti ingiusti e *ad personam*. Questa legge nasce infatti per vietare gli sconti di pena del rito abbreviato a chi si macchia di reati gravi puniti con l'ergastolo, e diventa una legge che serve ad allungare i processi a carico del Presidente del Consiglio per farli andare in prescrizione. Lo avete fatto come sempre con l'inganno, imponendo al Parlamento un voto di fiducia - l'ennesimo voto di fiducia - con la conseguenza di cambiare radicalmente il processo penale, ovviamente in peggio. Come è noto, noi dell'Unione di Centro e del Terzo Polo siamo sempre disponibili ad un confronto serio e di merito sulla riforma della giustizia ricordo che tra l'altro siamo in diretta televisiva. Mi farebbe piacere che si desse al Paese un'immagine più composta dei nostri lavori. in peggio. Come è noto, noi dell'Unione di Centro e del Terzo Polo siamo sempre disponibili ad un confronto serio e di merito sulla riforma della giustizia ovviamente se essa riguarda tutti i cittadini e non uno solo; se essa è funzionale alla concreta applicazione di principi e norme costituzionali, come il diritto di difesa ed il giusto processo; se la riforma si occupa di rendere più veloce ed efficiente il processo civile, creando così meccanismi virtuosi nelle relazioni economiche ed imprenditoriali. Purtroppo, oggi non ci stiamo occupando di questo, ma di un altro pasticcio, che come i precedenti è destinato ad impegnare inutilmente il Parlamento per finire al macero, come le altre leggi *ad personam*. Ci rifiutiamo infatti di pensare che questa legge sul "processo lungo" sia una cosa seria e che veramente voi la riteniate utile per il Paese. È infatti impossibile attribuire una qualsivoglia utilità sociale ad una legge che affida all'imputato il ruolo di regista esclusivo del suo processo: una legge che rende il giudice, il pubblico ministero e la vittima del reato inutili comparse. Siamo seri, cari colleghi: neanche voi pensate veramente di far approvare una legge che consente all'imputato di omicidio in una discoteca di citare come testimoni tutti coloro che erano presenti nel locale, obbligando il giudice a sentirli tutti, anche quelli che non sono in grado di fornire importanti elementi di prova. Neanche voi credete veramente che questa legge possa entrare in vigore, perché è oggettivamente inconcepibile che in un processo per omicidio, per violenza sessuale, per concussione, per sfruttamento della prostituzione l'imputato, per dimostrare di essere stato allo stadio il giorno in cui si è verificato il fatto, possa citare 3.000-4.000 tifosi che assistevano alla partita. Ci rifiutiamo di pensare che per voi il processo penale possa essere paralizzato da un capriccio dell'imputato. Ci rifiutiamo di pensare, onorevoli colleghi, che per voi il processo penale possa diventare un complesso sistema di scatole cinesi attraverso il quale riaprire processi diversi già conclusi con sentenze definitive, magari mettendo in discussione le decisioni assunte da altri magistrati perché non sono convenienti. Un processo così, onorevoli colleghi della maggioranza, non lo volete neanche voi, perché significherebbe seppellire principi fondamentali, come quello della certezza del diritto e quello della certezza della pena, di cui un tempo ormai lontano parlava anche la Lega Non possiamo pensare, cari colleghi della maggioranza, che introduciate norme così strampalate, che si devono applicare solo ad alcuni giudizi e non ad altri e che rischiano di far saltare il sistema della legislazione premiale per chi collabora con la giustizia e consente di colpire a morte la mafia e il terrorismo. Cari colleghi, non credo proprio che intendiate fare sul serio. Un tempo la vostra ossessione erano i pubblici ministeri; oggi, con questo provvedimento, diventa il giudice terzo chiamato a decidere. Non vorremmo che domani diventino gli avvocati che, anziché garantire il diritto di difesa come stabilisce la Costituzione, debbano operare nel giudizio secondo direttive vincolanti ed esclusive dell'imputato. Per questo motivo, vi diciamo no, perché quello che state approvando non è un provvedimento utile e serio, ma è solo un'altra perdita di tempo. Noi siamo interessati a parlare di riforme della giustizia, quelle vere, quelle che ci chiedono tutti (magistrati ed avvocati), quelle che dobbiamo scrivere insieme nell'interesse esclusivo del Paese, come anche ieri per l'ennesima volta il Capo dello Stato ci ha invitato a fare e voi non volete fare. Quando vi deciderete a fare le riforme per rendere efficiente la macchina della giustizia e per eliminare quelle oggettive storture che a volte compromettono seriamente i diritti fondamentali dei cittadini, noi saremo pronti come sempre a confrontarci. Da qui ad allora siamo interessati solo ad occuparci dei problemi veri del Paese, a cui non interessa proprio né il processo lungo né il processo breve. State, infatti, solo consumando una farsa. Per questo, vogliamo parlare di ciò che serve al Paese: noi vogliamo parlare del patto per la crescita, sottoscritto ieri da tutte le parti sociali, dal mondo delle banche a quello delle cooperative, dal sindacato agli imprenditori piccoli, medi e grandi, dagli agricoltori ai commercianti, agli artigiani. Un Governo responsabile, un Governo che ha a cuore l'Italia, nel momento più difficile per l'economia nazionale, non si occupa di cavilli legali o di scappatoie giudiziarie! Un Governo responsabile apre in Parlamento un confronto con le opposizioni, accogliendo l'appello delle parti sociali e l'invito del Capo dello Stato! Un Governo degno di questo nome si fa carico del documento unitario di tutte le categorie produttive del nostro Paese e fa proprie le loro preoccupazioni sull'andamento dei mercati finanziari, sulla debolezza dell'economia italiana, sulla fragilità istituzionale del contesto europeo in cui ci muoviamo, sulle preoccupazioni che derivano dalla crisi di bilancio degli Stati Uniti, sul pericolo che corre il nostro risparmio, quello delle famiglie italiane, che è il vero architrave del sistema nazionale. Un Governo intelligente avrebbe apprezzato la disponibilità delle opposizioni che hanno consentito una rapida approvazione della manovra economica per salvaguardare la credibilità internazionale dell'Italia e l'interesse nazionale. Un Governo che sente proprio il malessere economico e sociale degli italiani fa di tutto per evitare che le nostre famiglie ed i nostri figli debbano pagare debiti esosi che non hanno fatto e che non vogliono più fare! Noi vogliamo lavorare per il Paese, anche se siamo all'opposizione, e pretendiamo dal Governo che metta subito al primo punto della sua agenda, e di quella del Parlamento, il patto per la crescita. Pretendiamo da voi, colleghi della maggioranza, e dal vostro Presidente del Consiglio un vero atto di responsabilità, se ne siete capaci. Nel nostro Paese il disavanzo pubblico è al 4 per cento del prodotto interno lordo e il debito pubblico è vicino al 120 per cento del PIL. Sappiamo bene tutti che è necessario tagliare la spesa pubblica, ma il rigore dei conti deve essere funzionale - come giustamente dicono le parti sociali - alla crescita e allo sviluppo dell'economia. Se i tagli uniformi della spesa pubblica non innestano un circuito virtuoso di ripresa si rischia di sottrarre ossigeno all'economia italiana almeno per due punti del PIL in tre anni, come ci ricorda il governatore Draghi. Un'agenda per la crescita ha bisogno di decisioni rapide e spesse volte difficili, se si vogliono ridurre le tasse sui redditi dei lavoratori e delle famiglie e se si vuole fare una vera lotta all'evasione fiscale. Dall'avvio della ripresa ad oggi l'economia italiana ha recuperato solo due dei sette punti percentuali di PIL persi durante la crisi. Pensate, cari colleghi, che negli ultimi dieci anni il nostro prodotto è aumentato solo del 3 per cento a fronte del 12 per cento della Francia, che è un Paese simile al nostro. Il nostro Paese Paese attraversa una profonda crisi strutturale di produttività, e questa è omogenea, cari colleghi, dal Nord al Sud. Se la produttività ristagna, la nostra economia non può crescere, il sistema produttivo non è competitivo, si aprono dei disavanzi crescenti nella bilancia dei pagamenti e si inaridisce l'afflusso di investimenti diretti; calano le retribuzioni e calano i salari, e i consumi reali delle famiglie, che crescono (se crescono) solo erodendo il risparmio delle famiglie stesse. Per questi problemi gravi e seri, cari colleghi, ci vogliono Governi coraggiosi, risoluti e, soprattutto, umili; ci vuole una classe politica che sappia assumere decisioni impopolari. Di questo vogliamo parlare, di questo dobbiamo occuparci tutti insieme: non dei Ministeri al Nord, né di piccoli, ma devastanti interventi nel settore della giustizia. Questo dibattito è surreale, è lontano mille miglia dal Paese! Voltate pagina rapidamente se avete ancora un po' di rossore; occupiamoci dell'Italia, superando il profondo egoismo che occupa ancora Palazzo Chigi. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voteremo il disegno di legge Lussana che, lo dico senza tema di smentita, è stato oggetto in questi giorni di una vera e propria, scientifica campagna di disinformazione, in quest'Aula e fuori da quest'Aula. Abbiamo sentito dai colleghi dell'opposizione, anche da colleghi che dichiarano di essere esperti della materia processuale, delle vere e proprie menzogne, pronunciate senza alcun imbarazzo e con la sicurezza di chi sa che il giornalismo di questo strano Paese preferisce trincerarsi dietro qualche luogo comune che assurge a titolo di giornale, che fa vendere copie, piuttosto che fare la fatica di approfondire un provvedimento complesso, indubbiamente complesso, per informare correttamente i propri lettori. Innanzitutto, si è detto in quest'Aula che del progetto di legge presentato alla Camera dall'onorevole Carolina Lussana, e che riguarda la non applicazione di diminuzioni di pena nel caso di condanna all'ergastolo a seguito di rito abbreviato, non è rimasto nulla, e che ormai il provvedimento al nostro esame riguarda tutt'altro. Prima menzogna. Il progetto di legge Lussana, il cui *iter* è iniziato alla Camera nel giugno del 2010, conteneva un unico articolo che abrogava il secondo e terzo periodo del secondo comma dell'articolo 442 del codice di procedura penale. Ossia, il progetto di legge Lussana voleva che se il giudice condanna l'imputato all'esito del rito abbreviato all'ergastolo non dovesse esserci nessuna diminuzione di pena, come invece, purtroppo,

Poi, durante l'*iter* alla Camera, a quell'unico articolo del progetto Lussana ne sono stati aggiunti altri cinque, che avrebbero generato dei problemi di carattere processuale ed operativo evidenziati dall'Associazione nazionale magistrati.

442, chiarendo, al di là di ogni dubbio di qualsiasi azzeccagarbugli, che «quando, tenuto conto di tutte le circostanze, deve essere irrogata la pena dell'ergastolo, non si fa luogo alla diminuzione di pena». poi, in quest'Aula - seconda menzogna - che questo provvedimento è una schifezza, una fetecchia, una porcheria, un incubo e altri epiteti di questo tipo. Peccato che chi esprime questi giudizi non abbia letto l'articolo 111 della Costituzione, che contiene la stessa identica norma scritta in questo provvedimento. L'articolo

o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore». Il testo del nostro provvedimento

coraggio di dire che è una schifezza l'articolo 111 della Costituzione, che voi avete approvato nel 1999!

Oggi nell'articolo 190 del codice, che riguarda il diritto alla prova, si dice che il giudice ammette le prove dedotte dalle parti escludendo le prove vietate dalla legge e le prove manifestamente superflue o manifestamente irrilevanti: con la modifica proposta in questo provvedimento si dice che il giudice ammette le prove dedotte dalle parti escludendo le prove vietate dalla legge e le prove manifestamente non pertinenti. Ciò significa che il giudice deve ammettere le prove dedotte dalle parti (da tutte le parti, anche dai pubblici ministeri), non ammettendo le prove vietate dalla legge o le prove manifestamente non pertinenti al *thema decidendum*, con espressione più chiara più oggettiva e più corretta tecnicamente

alla seconda modifica. L'articolo 495 del codice di procedura penale sui provvedimenti del giudice in ordine alla prova dice che il giudice, sentite le parti - tutte le parti può revocare l'ammissione di prove che risultano superflue. Il provvedimento modifica questo articolo dicendo che il giudice, sentite le parti, tutte le parti, può revocare l'ammissione di prove che risultano superflue e manifestamente non pertinenti, salvo che siano state richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte.

- stabilisce che le sentenze irrevocabili di condanna possono essere acquisite come elemento di prova in un altro processo penale. Con questo provvedimento si

che tutta la dottrina ha chiesto al legislatore, sino ad oggi invano: ossia che, ferma restando la possibilità del giudice di acquisire come elemento probatorio a carico dell'imputato una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in un altro processo penale, deve rimanere fermo il diritto delle parti di ottenere l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza di condanna. Tuttavia, per scrupolo ulteriore, si è previsto che questa norma di civiltà che abbiamo aggiunto, che prevede l'esame delle persone, non si applichi comunque ai processi per reati di grave allarme sociale - quindi mafia, terrorismo e delitti sessuali - ossia quei delitti odiosi e gravissimi contenuti nell'articolo 51 del codice di procedura penale. Ricordatevi che la Corte costituzionale, quando ha salvato dalla incostituzionalità sicura questo articolo, in sostanza che quella sentenza di condanna pronunciata in un altro processo può valere come elemento probatorio a carico di un altro imputato, ma ha aggiunto che occorre avere elementi di conferma della sentenza, per rendere concreto ed effettivo il diritto al contraddittorio tra le parti nel momento della formazione della prova.

a favore di questo provvedimento, anche perché contiene due norme che modificano la legge Gozzini e che prevedono un severo sbarramento alla concessione dei benefici penitenziari per i condannati per delitti gravissimi.

*(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, il Paese attraversa la crisi più grave del dopoguerra; il Paese attraversa la crisi più grave dal dopoguerra. Quelli passati sono stati giorni molto intensi.

facendo lievitare i tassi di interesse dei nostri titoli pubblici, gravando di ulteriori gravi costi il nostro Paese e mettendo quindi in dubbio l'affidabilità sui mercati internazionali e nelle stesse relazioni internazionali,

assumendosi una parte di responsabilità che il Governo non era in grado, e non lo è ancora, di onorare. È esattamente di due giorni fa una posizione comune, per il tramite di un comunicato, di tutte le forze delle rappresentanze economiche e sociali del Paese, appello al quale pare non sia ancora giunta una risposta da parte del Ministro dell'economia, né tantomeno da parte del Presidente del Consiglio. forze economiche e sociali che, per dirla con la presidente Marcegaglia, si sentono abbandonate dal Governo e chiedono una discontinuità capace di realizzare un progetto di crescita, perché il rischio che la situazione diventi insostenibile è qui dinanzi a noi.

c'è da dire che a questo appello così solenne avrebbe dovuto opporsi ben altro che il provvedimento sul quale oggi il Governo pone la questione di fiducia. Non si arresta la tempesta sui mercati, e i nostri titoli pubblici sono ancora in grave situazione di crisi: e questo in un Paese nel quale il risultato delle elezioni, del *referendum* e degli stessi sondaggi

Il mio senso di responsabilità mi ha quindi impedito di dichiarare quello che penso». Dopodiché, vi è stata una sola conferenza stampa di illustrazione della riforma costituzionale, che non vedrà la luce in questa legislatura, per ragioni assolutamente legate alla cronologia dei lavori occasione dell'approvazione della manovra qui in Senato, si rispose dicendo che il presidente Berlusconi era scivolato su una saponetta; mi chiedo se stamattina si sia strozzato con il dentifricio.

per dire quali sacrifici sarà chiamato a fare, quali sono le prospettive e quali priorità verranno perseguite, per stare vicino all'Italia in questo momento difficile, sorreggerla e guidarla? La verità è che questo Paese non ha Presidente del Consiglio, né La prova conclamata sta nel fatto che oggi qui è stata posta la questione di fiducia su un provvedimento che si chiama processo lungo. Ora, collega Mazzatorta, alcune delle considerazioni che lei fa, non ci crederà, ma le condivido, solo che però sono solo parziali: probabilmente manca un pezzo, e magari sarebbe stato utile che noi ne discutessimo. Forse discutendone il pezzo sarebbe venuto compiuto in ogni sua parte, e la disposizione secondo cui l'imputato può interrogare o fare interrogare avrebbe avuto una norma di traduzione, perché così è il testo

Il problema è che i benefici arrivano quando la persona che si è resa colpevole di fatti gravi è già stata condannata, e già sta in carcere: il fatto è che se non ce la fate arrivare in carcere con una sentenza di condanna, non ci sarà mai beneficio che possa essere applicato applicato e durezza che possa essere invece usata! *(Applausi dal Gruppo PD)*. E voglio dirlo chiaro (io non adopero l'espressione che sempre viene adoperata), perché questa legge se può essere utile a qualcuno, se sarà utile a qualcuno, se deve essere approvata con il voto di fiducia per essere utile a qualcuno, e cioè al presidente Berlusconi, è un disastro per il resto. È un disastro per tutti quei cittadini che si aspettano una giustizia celere ed efficace: non avete mosso un dito su questo; siete stati capaci di creare meccanismi che renderanno assai più semplice commettere reati e farla franca. Detto questo, cari colleghi, mi pare ovvio che voteremo contro in questo voto di fiducia, e però voglio anche dire un'ultima cosa. Siccome io penso che fra di voi ce ne sono tanti, ma proprio tanti, che avvertono l'asprezza del momento e sentono cosa stanno chiedendo ai cittadini italiani, cosa sono costretti - loro ritengono - a chiedere, approvando provvedimenti economici che penalizzano le famiglie e le imprese (troppo duramente, secondo il nostro punto di vista), siccome molti di voi, come i colleghi della Lega,

loro e alla loro coscienza chiedo: era davvero così indispensabile che noi oggi fossimo chiamati ad un voto di fiducia non su una misura economica, non su una misura per la crescita, non per salvare le famiglie indigenti, non per aprire una prospettiva di lavoro ai ragazzi, non per dare una speranza speranza al Mezzogiorno, ma per approvare il "processo lungo"? Credo che quando sfilerete sotto quel banco

ed io non dubito che tra di voi molti sarebbero in grado di esserlo, molti sarebbero in grado di esprimere la loro di esprimere la loro natura di liberi e forti e di dare oggi all'Italia la prova che questo Governo è capace di badare ad altro che ad un *Premier* braccato che si chiude nelle sue stanze.

facoltà. GASPARRI *(PdL)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento che stiamo per votare è stato discusso qui a Palazzo Madama in seconda lettura. A quanti si sono indignati per i tempi, per il ricorso al voto di fiducia, sarà opportuno ricordare che questo provvedimento è stato approvato oltre tre mesi fa dalla Commissione giustizia ed è rimasto a lungo in lista di attesa prima di arrivare all'esame dell'Assemblea, senza alcuna fretta o forzatura. Ma nella Conferenza dei Capigruppo del 19 luglio - vi dà fastidio che noi lo si ricordi, ma è bene che anche l'opinione pubblica che ci segue e ci ascolta lo sappia - la calendarizzazione di questo provvedimento è avvenuta alla unanimità del parere dei Gruppi parlamentari. Quindi, nessuna forzatura! Quando siamo arrivati in Aula sono state presentate 11 o 12 questioni pregiudiziali ed altre - per carità, legittime perché previste dal Regolamento - iniziative di carattere ostruzionistico, così come quando il relatore Centaro - che ringrazio, come ringrazio il capogruppo Mugnai e tutti i colleghi che hanno lavorato in questi mesi con il presidente Berselli ed altri senatori a questo provvedimento - ha presentato un emendamento che andava in una direzione ancora più restrittiva nel rispetto del principio della certezza della pena che questa legge garantisce ampiamente, come hanno già detto i colleghi Mazzatorta, Centaro ed altri, e voi avete presentato 70 subemendamenti, con un chiaro intento ostruzionistico, che rende legittimo il voto di fiducia. Voi potete fare la vostra opposizione, noi abbiamo diritto di portare all'approvazione una legge in cui crediamo. Avete alimentato di bugie questa fase di discussione; giornali che hanno scritto: ci sarà l'emendamento "blocca-Ruby", ci saranno norme che favoriscono la mafia. Avete alimentato la macchina delle bugie di fronte a fatti inesistenti e ad emendamenti mai pensati e mai e Belisario).* Per quanto riguarda, senatore Li Gotti, il capitolo antimafia, gli emendamenti che le citava li ha presentati il senatore Mugnai. Questa norma non condiziona in alcun modo i processi contro la mafia e la criminalità organizzata che non subiranno alcun rallentamento e rivendichiamo alla maggioranza una volta di più l'impegno che abbiamo rispettato di varare in questa legislatura le più severe leggi antimafia. Siamo stati noi a dar luogo ad una legislazione *(Applausi dal Gruppo PdL)* a fronte di presunte icone della Repubblica - ne rifaccio il nome ancora una volta - come Ciampi, Scalfaro, Amato e Mancino che guidavano le istituzioni quando il carcere duro, il 41-*bis*, veniva cancellato per centinaia di appartenenti alle cosche.

Colleghi, togliete quei cartelli, immediatamente! Non siamo qui per fare degli *show*. Ne terrò conto in occasione della prossima richiesta di diretta televisiva da parte del Gruppo dell'Italia dei Valori. Ne terremo debitamente conto. Togliete quei cartelli. Ne terrò conto. Senatore Pedica! *(Gli Ne terremo debitamente conto quando chiederete nuovamente una diretta televisiva. Continui, presidente Gasparri. c'è qualcuno che quando si ricorda che altri hanno cancellato il carcere duro cerca di impedire di affermare la verità. Ma noi affermeremo la verità in quest'Aula ed ovunque *(Applausi dal Gruppo PDL)* nonostante che per alcuni, con il piede di qualche altro padrone a cui si ispira, scatti la molla. Questa legge applica il principio del nuovo articolo 111 della Costituzione, articolo che fu approvato quando era ministro della giustizia - pensate un po' - Oliviero Diliberto. Quindi credo che questo riferimento ad un esponente della della sinistra, di quella più estrema, ricordi che quell'atto fu condiviso ampiamente dal Parlamento. Quindi, portiamo questi principi per un giusto processo all'interno di questa legge. Abbiamo anche introdotto, con questa normativa, Abbiamo anche introdotto, con questa normativa, dei principi che garantiscono che i reati puniti con l'ergastolo non avranno riduzioni e per i delitti più efferati non ci saranno più benefici penitenziari. Quindi gli italiani hanno oggi una legge, approvata dal Senato, che garantisce di più la gente onesta nei confronti Per quanto riguarda altri aspetti, noi riteniamo che sia giusto affermare anche altri principi di diritto. Le sentenze passate in giudicato producono fonte di prova. Però noi riteniamo che chi è stato estraneo ad altri giudizi debba poter verificare le accuse contro di lui. È un principio di civiltà giuridica. Si è parlato di regime; ma il vero regime sarebbe quello in cui un imputato debba subire l'applicazione di una sentenza di un processo al quale non ha partecipato. I principi ingiusti non saranno mantenuti solo perché li volete utilizzare voi *ad personam* contro chi volete distruggere attraverso un uso politico della giustizia.

può essere santificata, se serve a proseguire con altri mezzi una battaglia di natura politica. Quindi i principi ingiusti non debbono essere mantenuti. il rispetto dell'articolo 111 della Costituzione, la possibilità di una discussione paritaria tra le parti nel processo. E non ci saranno allungamenti indefiniti dei processi; così come i processi contro la criminalità potranno proseguire con speditezza - e in questo dibattito sono emerse con chiarezza le menzogne che avete detto - e i giudici potranno cancellare dalle liste di testimoni inserimenti pretestuosamente realizzati. Quindi la ragionevole durata del processo sarà garantita anche da questa norma. È inutile che alimentiate, con la disinformazione e con la macchina delle bugie, la vostra campagna politica. Noi riteniamo che il voto di fiducia sia più che giustificato di fronte all'ostruzionismo. E proseguiremo in un'azione di riforme: riforme costituzionali della giustizia e riforme costituzionali del Parlamento e del Governo, che approveremo in questa legislatura, così come abbiamo affrontato i temi dell'economia. Diamo atto al Parlamento di aver avuto momenti di responsabilità, quando si è varata nei giorni scorsi la manovra; ma non accettiamo richiami. Abbiamo varato provvedimenti sullo sviluppo e stiamo affrontando una difficile situazione economica, dove le borse europee e quella italiana risentono ogni giorno di quel che accade in Grecia e negli Stati Uniti. Stiamo seguendo, come se fosse una vicenda italiana, la trattativa tra democratici e repubblicani americani, perché da essa dipende anche l'andamento delle economie europee, l'attacco all'euro e le speculazioni. È un dovere civile difendere l'interesse nazionale, non è certo una vostra concessione difendere i diritti degli italiani, la nostra economia, la nostra Nazione! *(Applausi dal Gruppo PdL).* E noi, come hanno ricordato ieri alcuni colleghi, lo abbiamo fatto, quando voi al Governo non avevate i numeri per sostenere una politica internazionale e missioni militari all'estero. Noi avevamo la maggioranza e vi diamo atto di atteggiamenti responsabili. Ancor più lo siamo stati noi, quando non avevate i numeri per difendere il buon nome dell'Italia nel mondo; e noi siamo stati presenti e responsabili! concludo, signor Presidente - non c'è nessun piede del padrone e non c'è nessun regime. Noi facciamo liberamente una legge giusta. Voglio dire a chi parla, quasi con una sorta di innato senso di superiorità morale, che se un regime c'è, senatore Zanda, lo vada a cercare a Sesto San Giovanni, dove da padre in figlio i sindaci alimentano un sistema di illegalità, che riguarda la vostra della senatrice Bassoli).* Questo è il regime, laddove imprese, cooperative, territori, gestione globale hanno dimostrato come qualcuno si è impossessato di pezzi d'Italia. Se cercate il regime, non avete bisogno di andare lontano. Guardatevi Guardatevi allo specchio e lo troverete nel vostro passato e nel vostro presente.

abbinare la severità nei confronti di chi commette crimini con il diritto pieno di ogni cittadino di fronte alla giustizia. Questa è la nostra posizione e la difendiamo con convinzione, non accettando lezioni di moralità da parte di chi non ha titolo per impartirne.

Colleghi, prima di passare al voto, vorrei ricordare che l'Aula tornerà a riunirsi lunedì prossimo, alle ore 17, per discutere il bilancio interno del Senato. Durante tale seduta saranno anche possibili votazioni.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. *(È

Caruso,

D'Ambrosio

Ai fini del verbale, diamo atto che a votazione chiusa la senatrice Carlino è arrivata in Aula, ma non ha potuto partecipare al voto in quanto era già in corso il computo dei